per favore,

Comunico di avere ricevuto la seguente lettera: «Roma, 7 dicembre 2016 Onorevole Presidente, La informo che in data odierna ho rassegnato al Capo dello Stato le mie dimissioni. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a restare in carica per il disbrigo degli affari correnti. *F.to* Matteo Renzi».

La informo che il Presidente della Repubblica, con propri decreti in data 12 dicembre 2016, ha accettato le dimissioni rassegnate il 7 dicembre 2016 dal Gabinetto presieduto dal dottor Matteo RENZI, nonché le dimissioni dalle rispettive cariche rassegnate dai Sottosegretari di Stato. Avendo accettato l'incarico di formare il Governo conferitomi in data 11 dicembre 2016, il Presidente della Repubblica mi ha nominato, con proprio decreto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

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il dottor Gian Luca GALLETTI; - delle Infrastrutture e dei trasporti, il dottor Graziano DELRIO; - del Lavoro e delle politiche sociali, il signor Giuliano POLETTI;

Inoltre, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 12 dicembre 2016 adottato su mia proposta e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato l'onorevole avvocato Maria Elena BOSCHI Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo».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 alla dott.ssa Anna FINOCCHIARO i rapporti con il Parlamento; - all'onorevole dottoressa Maria Anna MADIA la semplificazione e la pubblica amministrazione; - all'on. dott. Enrico COSTA gli affari regionali;

sta rendendo le proprie dichiarazioni programmatiche presso la Camera dei deputati. La consegna del testo al Senato avrà luogo intorno alle ore 12,30. Successivamente la seduta sarà sospesa e verrà ripresa per comunicare le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo che si riunirà alle 15,30. prima di sospendere la seduta, saluto la delegazione della formazione umanitaria FAC del Senegal che assiste ai nostri lavori.

Presidente, onorevoli senatori, consegno il testo delle dichiarazioni rese stamani alla Camera dei deputati, sulle quali svolgeremo domani il dibattito. Grazie e buon lavoro. Ringrazio il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Gentiloni Silveri, e prendo atto della consegna del testo delle dichiarazioni programmatiche già rese alla Camera dei deputati.

finestra"). Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha definito l'organizzazione del dibattito sulla fiducia al Governo. La discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgerà nella seduta unica di domani, con inizio alle ore 9,30. Per la discussione sono state ripartite 3 ore e 15 minuti sulla base di specifiche richieste dei Gruppi. La replica del Presidente del Consiglio dei ministri, prevista per le ore 13, e le successive dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno luogo con trasmissione diretta televisiva. La chiama avrà inizio intorno alle ore 15.

discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgerà nella

Grazie